Fermi restando i disegni di legge e gli altri argomenti già previsti dal calendario corrente, è stato stabilito che nella seduta pomeridiana di mercoledì 25 novembre, a partire dalle ore 16,30, saranno discusse le mozioni Zanda e Belisario concernenti il sottosegretario Nicola Cosentino. I Gruppi avranno complessivamente a disposizione 18 minuti ciascuno. La data della seduta riservata allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, al momento prevista per il pomeriggio di giovedì 26 novembre, potrebbe subire variazioni in relazione alla disponibilità dei Ministri. Nella seduta pomeridiana di martedì 1° dicembre la Presidenza ricorderà la figura di Luigi Granelli a dieci anni dalla sua scomparsa. I rappresentanti dei Gruppi potranno intervenire per 5 minuti ciascuno. Nella seduta pomeridiana di mercoledì 2 dicembre, con inizio alle ore 16,30, saranno poste all'ordine del giorno mozioni sulle riforme costituzionali. I Gruppi avranno complessivamente a disposizione 20 minuti ciascuno. Dopo la festività dell'8 dicembre, l'Assemblea tornerà a riunirsi nella seduta pomeridiana di mercoledì 9 e nella seduta antimeridiana di giovedì 10 per la discussione di mozioni i cui argomenti saranno successivamente definiti. Nel pomeriggio di giovedì 10 dicembre, alle ore 15, avrà luogo il sindacato ispettivo. Infine, la Presidenza ha proceduto a una nuova ripartizione dei tempi di esame del disegno di legge collegato in materia di lavoro pubblico e privato,

commi 2 e 3 del decreto ministeriale n. 270 del 2004, rientra nell'autonomia degli atenei attivare e/o disattivare i corsi di studio, si comunica che il problema sollevato dai senatori interroganti è stato superato. Infatti, in merito al corso di laurea magistrale in informazione e sistemi editoriali, già attivato presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», con il decreto rettoriale n. 2102 del 15 giugno 2009, rilevata la sussistenza dei requisiti minimi previsti dalla vigente normativa, è stato disposto l'inserimento del corso medesimo nell'ambito dell'offerta formativa dell'anno accademico 2009-2010, per il quale sono regolarmente aperte le iscrizioni. Signor Presidente, ringrazio il Sottosegretario. Presumo che il collega Pardi aggiungerà qualche altra considerazione, perché sua omologa interrogazione è a testimoniare la preoccupazione che in quel frangente si determinò nel mondo degli insegnanti e degli studenti per il rischio di chiusura di una delle attività

un rischio che rimane immanente, signor Sottosegretario, perché i tagli così virulenti apportati all'università fanno sì che tanti corsi di laurea siano legati a delle contingenze piuttosto che a delle strategie formative.

quanto un impegno affinché questa parte rilevante dell'attività formativa non venga ingoiata da una politica di tagli e di riduzione

degli ultimi decenni è proprio la proliferazione, qualche volta francamente assai discutibile, sia delle sedi che dei corsi di laurea. Noi, in questo caso, ci eravamo mossi perché

occorre fare lo sforzo analitico e scientifico di individuarli. Se invece ci si trova di fronte a un corso seguitissimo dagli studenti, anche con un certo entusiasmo, appoggiato dal rettore, nonché da un'opinione pubblica scientifica rispettabile, è chiaro che la situazione è non si riproponga il prossimo anno. Siamo invece disponibili in futuro, quando si presenterà l'occasione, a discutere della dimensione universitaria, con una saggezza che forse, nel passato, è stata un po' carente.

Presidente, premetto che la circolare n. 38 del Ministero del 2 aprile 2009, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto interministeriale riguardante le dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2009-2010, al paragrafo «Istruzione secondaria di II grado» prevede che il numero delle classi prime venga determinato tenendo conto del numero complessivo degli alunni, indipendentemente dalla distribuzione degli stessi tra i diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento. Nelle operazioni di definizione dell'organico di diritto, la fase istruttoria consente alle istituzioni scolastiche e all'ufficio scolastico territoriale di determinare l'organico attraverso un confronto inteso a raggiungere l'obiettivo di una più razionale distribuzione delle risorse, nel rispetto delle dotazioni organiche assegnate agli uffici scolastici regionali. In merito al caso evidenziato dall'onorevole interrogante, riguardante l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato «Cine TV Rossellini» di Roma, il competente direttore dell'ufficio scolastico regionale del Lazio ha fatto presente che, in data 20 marzo 2009, il dirigente scolastico dell'istituto in questione ha inviato una proposta di organico, relativa all'anno scolastico 2009-10, per la formazione di otto classi prime con un numero complessivo di 166 alunni di cui quattro alunni disabili. La suddetta richiesta prevedeva la costituzione di sei classi prime dell'indirizzo AC (biennio audiovisivo, con 133 alunni di cui due disabili), una classe prima dell'indirizzo AF (biennio fotografia, con 18 alunni di cui un disabile, a fronte di 17 richieste di iscrizione), ed una classe prima dell'indirizzo UZ (biennio grafica pubblicitaria, con 15 alunni di cui un disabile). Non ricorrendo i presupposti per la costituzione di classi prime per tutti gli indirizzi di studio richiesti dal dirigente scolastico, nella fase istruttoria l'ufficio scolastico provinciale ha comunicato al dirigente medesimo, in data 15 aprile 2009, la modifica di tale proposta, non autorizzando le prime classi degli indirizzi biennio fotografia e biennio grafica pubblicitaria, in quanto il numero degli allievi iscritti non risultavano rispondenti ai parametri stabiliti dalla normativa vigente. Successivamente, alla luce di quanto rappresentato dal dirigente scolastico in data 17 aprile 2009, l'ufficio scolastico territoriale, compatibilmente con le risorse assegnate, ha accolto parzialmente le richieste del dirigente scolastico, autorizzando l'indirizzo del biennio fotografia (AF), in considerazione dell'unicità dell'indirizzo sul territorio. Il medesimo dirigente dell'ufficio scolastico regionale, nonostante ogni migliore determinazione, non ha invece potuto accogliere la richiesta di attivazione dell'indirizzo UZ biennio grafica pubblicitaria - considerato l'esiguo numero di alunni (15) rispetto ai parametri numerici stabiliti dalla vigente normativa. Infatti, mentre per l'indirizzo AF biennio fotografia - ricorrono le condizioni previste dalla circolare ministeriale n. 38 (unicità sul territorio e salvaguardia del corso unico), tali da giustificare la costituzione di una classe sottodimensionata, per l'indirizzo UZ -biennio grafica pubblicitaria - non si sono ravvisate tali condizioni, in quanto sul territorio, in ambito provinciale e comunale, esistono nove istituzioni scolastiche presso le quali sono state autorizzate classi di detto indirizzo presenti anche nei distretti scolastici 17 e 21, viciniori all'Istituto professionale in questione.

risposta. Vorrei svolgere alcune precisazioni. Certamente siamo consapevoli della rigidità della normativa, ma siamo anche consapevoli (e penso che in qualche modo questa attenzione vi sia stata nel definire poi la possibilità che ci fosse il percorso di fotografia, per quello che riguarda la scuola Rossellini) della necessità di aggiungere il buon senso rispetto a quelle che sono le più rigide normative. Il Sottosegretario ha già detto che in questo caso c'è l'unicità nel Lazio di questa specialità che, peraltro, ha una valenza particolare, perché abbiamo qui delle scuole di formazione professionale di alta qualificazione, che in realtà consentono poi ai ragazzi di trovare lavoro, fino ad oggi così è successo. È chiaro che dobbiamo, io credo tutti insieme, avere particolare attenzione a sostenere quelle realtà scolastiche che non solo qualificano i nostri giovani, ma consentono loro successivamente di trovare uno sbocco professionale autonomo. Comprendo anche la riflessione che il Sottosegretario ha posto rispetto alla non unicità del percorso della grafica. Si potrebbe fare successivamente un passo avanti. Dalle cose che il Sottosegretario ha detto e da quello che ho potuto sapere, si è parlato di un'attivazione per quest'anno, facendo riferimento all'organico di fatto e quindi lasciando il percorso incerto per questo corso che abbiamo detto essere così significativo rispetto alla sua unicità. Ci auguriamo che il passo successivo possa essere quello di stabilizzare questa realtà perfezionando il passaggio dall'organico di fatto all'organico di diritto, perché credo sia interesse comune

attribuisce all'Agenzia stessa il compito di sottoporre al Ministero il Piano aerospaziale nazionale (PASN) con valenza triennale, si fa presente che il Piano 2009-2011, che identifica gli obiettivi di breve-medio periodo nel solco di una più ampia strategia di lungo termine, è stato già approvato dal nuovo consiglio di amministrazione. Il Ministero, quindi, a valle delle opportune consultazioni con la comunità scientifica, l'industria, i centri di ricerca nazionali e le altre amministrazioni dello Stato competenti, procederà agli adempimenti formali per l'approvazione del Piano medesimo. Si concorda con il senatore Latronico, che evidenzia il rilievo nazionale ed internazionale del Centro di geodesia spaziale «Giuseppe Colombo» di Matera, una delle principali strutture di ricerca del Mezzogiorno che nel tempo ha incrementato le sue competenze ed oggi ospita attività gestionali, operative e formative nelle discipline di geodesia spaziale, telerilevamento e robotica spaziale; è, inoltre, fornita di un'imponente e innovativa dotazione di infrastrutture e di personale con elevate competenze scientifiche ed ospita tutte le attività operative di osservazione della terra dell'Agenzia spaziale italiana: in particolare, presso il Centro è operativo lo *User Ground Segment* civile della Missione Cosmo-SkyMed, responsabile dell'acquisizione, del processamento e della distribuzione dei dati rilevati per applicazioni civili. Il Centro rappresenta una delle poche stazioni fondamentali della rete mondiale di geodesia spaziale, poiché ospita con tecnologia allo stato dell'arte le tre tecniche osservative fondamentali (SRL/LLR, VLBI, GPS) oltre ad un gravimetro assoluto di altissima precisione; va anche ricordato che in Europa sono presenti solo due stazioni di tale tipologia: il nostro centro e la stazione tedesca di Wettzell. Per quanto riguarda la verifica dell'opportunità di istituire presso il Centro di Matera un dipartimento con funzioni di coordinamento e gestione dell'attività di ricerca sia nel campo geodetico che in quello del telerilevamento, si fa presente come il Centro medesimo già rappresenti il punto di riferimento riconosciuto a livello nazionale ed internazionale per le reti geodetiche e per le attività operative di telerilevamento. oltre alle funzioni per la missione Cosmo-SkyMed, il Centro è l'unica struttura nazionale che elabora dati satellitari delle missioni di osservazione della terra dell'Agenzia spaziale europea. Va sottolineato che il compito istituzionale dell'Agenzia spaziale italiana è quello di promuovere e supportare l'attività scientifica mettendo a disposizione gli *asset* spaziali di cui è responsabile e curando il raccordo con gli istituti scientifici utilizzatori; in particolare, il Centro di Matera già efficacemente gestisce il coordinamento con gli istituti scientifici demandati alle scienze geodetiche e di telerilevamento. A conferma che la valorizzazione del Centro è alla costante attenzione dell'ASI e del Ministero, si riferisce, infine, che proprio lo scorso martedì 17 è stato firmato un accordo tra ASI e la Regione Basilicata

lo scopo di ribadire l'interesse nazionale verso questa struttura che nel tempo, come riconosceva nella risposta all'interrogazione il Governo, ha guadagnato un'importante presenza di competenze e di impiantistica, necessarie a gestire nella rete mondiale delle osservazioni il tema del telerilevamento e del settore geodetico in generale.

scongiurare che si viva di un passato mentre magari il presente sfugga ad alcune certezze. Mi riferisco, in particolare, al protocollo d'intesa cui lei faceva riferimento, su cui vorrei fare alcune osservazioni. Dobbiamo evitare che il protocollo d'intesa resti tale, perché la sua attuazione è demandata ad un accordo di programma che dovrebbe concretizzare la collaborazione tra l'ASI, che impiega un certo*budget* di risorse, e la Regione Basilicata. momento, infatti, non vi è traccia di risorse, né nei bilanci dell'Agenzia spaziale italiana, né, per la verità, in quelli della Regione Basilicata, che si impegna a produrre le necessarie variazioni. Dobbiamo poi scongiurare

piccole e medie imprese locali, che in questi anni faticosamente sono nate attorno al Centro di geodesia. Dobbiamo quindi far sì che tali investimenti tecnologici importanti, questo capitale di cui abbiamo parlato, produca anche l'attrazione di investimenti industriali ad alta tecnologia. In una parola, signor Sottosegretario, dobbiamo evitare, e su questo continueremo ad esercitare la nostra vigilanza, che il Centro di Matera sia una grande commessa esclusivamente o prevalentemente per Finmeccanica ed il mondo che gira attorno a questa società, affinché il reticolo delle piccole e medie imprese cresciute in questi anni che stanno dando vita ad un sorta di distretto tecnologico interno a Telespazio e al Centro di geodesia spaziale possa prendere corpo nel tempo. Per quanto ci riguarda, continueremo a vigilare affinché tali obiettivi si realizzino davvero.

Signor Presidente, con riferimento all'interrogazione presentata dal senatore Li Gotti, concernente la richiesta di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato per il dottor Emilio Brogi, si rappresenta

di due professionisti del libero foro. Il Dicastero della giustizia ha riferito, in merito, che la procura della Repubblica di Catanzaro Direzione distrettuale antimafia ha fatto presente che Emilio Brogi e Aldo Cosentino sono imputati di concorso in corruzione aggravata (articoli 318, 319 e 321 del codice penale

ha precisato che l'imputato Brogi non è difeso dall'Avvocatura dello Stato, mentre 1'imputato Aldo Cosentino, nella qualità di direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è difeso dall'Avvocatura dall'Avvocatura dello Stato di Catanzaro. L'Avvocatura generale dello Stato fa conoscere che non corrisponde al vero la notizia, fornita da organi di stampa, secondo la quale la stessa Avvocatura avrebbe assunto il patrocinio del dottor Emilio Brogi nell'ambito dell'indagine, denominata «Perseus», condotta dai sostituti procuratori della Direzione distrettuale antimafia presso la procura della Repubblica di Catanzaro. Fa presente, altresì, che, nell'ambito del medesimo procedimento penale, il direttore generale della Direzione per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente, dottor Aldo Cosentino, imputato dei reati di cui agli articoli 81,110, 318, 319, 321 del codice penale e 7 della legge n. 203 del 1991, si è avvalso della facoltà di chiedere il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 44 del regio decreto n. 1611 del 1933. La richiesta di patrocinio, accompagnata dal parere favorevole del Ministro dell'ambiente, è stata accolta dall'Avvocato generale dello Stato con nota protocollo n. 84154 del 12 marzo 2009, essendosi valutato, sulla base di un esame degli atti, che la difesa nel giudizio penale del direttore generale del Ministero dell'ambiente fosse coincidente con l'interesse pubblico a ribadire, al tempo stesso, la legittimità dell'operato dell'amministrazione nel procedimento relativo alla classificazione come zona di protezione speciale dell'area su cui sarebbe dovuto sorgere il complesso turistico-residenziale Europaradiso. L'Avvocatura generale dello Stato, infine, comunica che, nell'udienza del 19 ottobre ultimo scorso, di discussione della posizione del dottor Aldo Cosentino, è stata chiesta l'assoluzione dell'imputato con formula piena *ex* articolo 530, primo comma, del codice di procedura penale e che l'udienza per le eventuali repliche dell'accusa è fissata per il 26 novembre 2009.

Signor Sottosegretario, apprendiamo così che ci sarebbe una convergenza con la finalità pubblica svolta nell'interesse dello Stato da parte dell'Avvocatura nella difesa di un imputato per corruzione in atti contrari ai doveri d'ufficio aggravata dalla finalità mafiosa, per una vicenda che vede coinvolto un gran numero di imputati e che riguarda la realizzazione sulla carta di un insediamento turistico su un'area di 1.000 ettari con un investimento di 7 miliardi di euro,

che quella zona a protezione speciale doveva essere così classificata in Europa, sennonché, secondo l'accusa, il direttore generale del Ministero Cosentino aveva fatto in modo di non far pervenire alle autorità europee la documentazione per non far inserire quest'area fra le zone a protezione speciale, così consentendo la realizzazione di quel megaprogetto. Il fatto che la difesa abbia assunto, nella sua discussione avvenuta negli scorsi giorni, l'insussistenza dell'addebito nulla toglie al fatto che il pubblico il pubblico dipendente è imputato di fatti aggravati dalla condotta mafiosa unitamente a capi di organizzazione mafiosa, dei clan ben noti. Mi lascia francamente stupito come possa ritenersi coincidente con la finalità pubblica un ruolo che secondo un'accusa - e c'è un processo in corso - vede lo Stato parte danneggiata. Qui lo Stato invece è coinvolto, attraverso gli organi della pubblica accusa e i pubblici Ministeri della procura antimafia, a sostenere la condanna del pubblico dipendente e gli avvocati dello Stato, organi dello Stato, a sostenere la difesa, mentre in quel processo lo Stato doveva costituirsi parte civile.

il Comune di Rubiera, con nota del 19 luglio del 2005, a valle degli approfondimenti effettuati relativamente alle opere di viabilità da realizzare a cura di TAV (società controllata da RFI per la progettazione e la costruzione delle linee ferroviarie veloci) ed in ottemperanza agli accordi sottoscritti nella Conferenza dei servizi del 31 luglio del 1998, richiesto di non procedere con la realizzazione del sottopasso di via del Benefizio evidenziando l'opportunità di realizzare, in sostituzione del suddetto sottopasso, nuovi interventi di viabilità finalizzati ad alleggerire gli impatti dovuti alla realizzazione delle opere AV/AC in aree già fortemente penalizzate dai transiti veicolari. Tali interventi alternativi sono stati individuati dall'amministrazione comunale e consistono nella realizzazione di un ponte sul torrente Tresinaro, con relativi raccordi stradali, per congiungere la Strada provinciale 51 a via delle Chiuse, e di un tratto di pista ciclopedonale tra l'abitato di San Faustino e Rubiera. A seguito di tale richiesta, accolta da TAV a condizione di mantenere invariato il quadro economico complessivo degli interventi, è stato sottoscritto in data 3 agosto 2005 tra il Comune di Rubiera, la Provincia di Reggio Emilia, TAV il consorzio Cepav Uno un accordo modificativo ed integrativo dell'accordo integrativo e della convenzione sottoscritti il 31 luglio del 1998, per disciplinare le modalità di attuazione dei nuovi interventi. L'accordo, approvato dal consiglio comunale di Rubiera il 7 luglio del 2005 e dalla giunta provinciale di Reggio Emilia il 5 luglio del 2005, stabilisce che TAV, tramite Cepav Uno, in sostituzione delle obbligazioni relative alla realizzazione del sottopasso di via del Benefizio, proceda alla realizzazione del ponte sul Tresinaro e dei relativi collegamenti con la viabilità esistente (opere concluse e attive dal marzo del 2009) e che il Comune di Rubiera realizzi direttamente un tratto di circa 2 chilometri di pista ciclopedonale tra la frazione di San Faustino e l'abitato di Rubiera, con un contributo di TAV completato nel 2008 con l'erogazione del contributo di 1,6 milioni di euro. Inoltre, al momento della stipula del suddetto accordo, erano in corso di realizzazione alcune solette ed elevazioni delle rampe del sottopasso di via del Benefizio. Tali opere, oggi demolite, corrispondono a circa il 5 per cento dell'intero intervento di via del Benefizio, che era costituito, oltre che dalle strutture delle stesse rampe, dal sottopasso ferroviario AV, dal sottopasso autostradale, dalle opere di finitura nonché dagli allargamenti autostradali.

poneva domande un po' diverse rispetto alla risposta del Sottosegretario. La questione è questa: per la realizzazione dei lavori della TAV è stato demolito un ponte sopraelevato che attraversava una carreggiata autostradale lungo via del Benefizio, un'antica e prestigiosa strada che si trova nel territorio comunale di Rubiera. La TAV aveva stanziato 4,5 milioni di euro per la costruzione di alcune infrastrutture della zona, in particolare un sottopasso che doveva garantire l'accesso ai poderi che erano rimasti isolati a causa della demolizione del ponte. Questa è la questione: se si demolisce un ponte si deve fare un sottopasso. È successo che la realizzazione del sottopasso è iniziata regolarmente dopo che erano stati espropriati e occupati di urgenza terreni e porzioni di aree al fine di predisporre i lavori per la TAV, ma dopo che è stata iniziata l'opera

che era già costata 700 milioni di euro, cui vanno aggiunti 500 milioni per i costi di lavorazione, è necessaria per permettere agli agricoltori della zona di raggiungere i poderi: questi infatti sono rimasti isolati e chi vuole accedervi deve immettersi sulla strada provinciale e allungare notevolmente il

indispensabili anche in considerazione dei denari pubblici spesi. In secondo luogo si chiedeva se non si intendesse effettuare un'indagine approfondita

nella galleria di Seiano, in Comune di Vico Equense in conseguenza dei lavori di adeguamento della variante alla statale Sorrentina, l'ANAS Spa ha fatto conoscere che il progetto di tali lavori prevede un'unica galleria di collegamento tra le località Pozzano, nel territorio di Castellammare di Stabia e Seiano, nel territorio di Vico Equense, includendo l'attuale galleria in esercizio che bypassa l'abitato di Vico Equense (galleria di Seiano). Per realizzare la continuità delle complesse opere civili di innesto tra la galleria in costruzione e quella esistente, consentire l'esecuzione delle piazzole di sosta in galleria, l'esecuzione del canale di ventilazione e degli impianti tecnologici (impianto di illuminazione, antincendio e sistemi di sicurezza) all'interno dell'attuale galleria di Seiano occorre necessariamente interdire al transito la galleria deviando obbligatoriamente il traffico veicolare lungo il vecchio percorso della strada strada statale 145 Sorrentina che attraversa il centro cittadino di Vico Equense. A questo fine, l'ANAS ha istituito, sin dal novembre 2007, un tavolo di concertazione con tutti i soggetti, le associazioni e gli enti territorialmente coinvolti (Ministero delle infrastrutture e trasporti, Regione Campania, amministrazioni comunale, Polizia stradale, circumvesuviana, associazione degli albergatori). In tale ambito, è emersa la decisione di prevedere la chiusura della galleria di Seiano a decorrere dal mese di ottobre 2008. Per quanto concerne la durata dei lavori previsti all'interno della galleria di Seiano, questi sono ripresi il 22 ottobre ultimo scorso, secondo il cronoprogramma allegato alla perizia di variante tecnica. Il termine di ultimazione dei lavori è previsto al 15 aprile 2011. La perizia concerne l'adeguamento dell'opera agli standard di sicurezza previsti dal nuovo quadro normativo in materia di circolazione stradale in galleria. Inoltre, è stato previsto un ingresso intermedio in galleria, utilizzando un tratto della vecchia galleria Seiano, al fine di creare un *by-pass* alla nuova galleria per evitare l'interessamento, l'interessamento, nel caso di incidente o di traffico intenso, del centro abitato di Vico Equense. Tra le altre iniziative per la soluzione delle problematiche viabilistiche, si menziona la sottoscrizione di un'apposita convenzione tra ANAS e le amministrazioni comunali della Penisola sorrentina, dell'importo complessivo pari a 600.000 euro, finalizzata al potenziamento dei servizi di polizia stradale lungo il percorso alternativo che il traffico veicolare è costretto a seguire nell'interno dell'abitato di Vico Equense. Al fine, poi, di ridurre i disagi alla mobilità da e per la Penisola sorrentina, la giunta regionale della Campania, su proposta dell'assessore ai trasporti, ha approvato un finanziamento di 1.300.000 euro per il potenziamento delle vie del mare lungo la direttrice Napoli-Castellammare di Stabia-Sorrento.

ulteriore pregiudizio al completamento dei lavori per la mancata e/o ritardata chiusura della galleria di Seiano. In tale ambito, dopo ampia discussione ed in considerazione delle istanze esposte dai rappresentati del territorio, sono state condivise le tre finestre temporali (dall'8 gennaio 2009 al 31 marzo 2009; dal 15 ottobre 2009 al 15 aprile 2010; dal 15 ottobre 2010 al 15 aprile 2011) citate dell'interrogante all'interno delle quali la galleria sarà completamente chiusa per consentire di proseguire utilmente le lavorazioni su tre turni lavorativi. Durante la prima finestra temporale di chiusura (8 gennaio - 31 marzo 2009) si è potuto registrare, a meno di sporadici episodi, un rallentamento del flusso veicolare diretto da e per Sorrento, con allungamento del tempo medio di percorrenza, nelle ore di massimo afflusso, valutato in circa quindici L'ANAS ha fatto tuttavia conoscere che l'approvazione della perizia di variante tecnica ha consentito di modificare il secondo periodo di chiusura della galleria, che è stato variato dal 22 ottobre 2009 al 31 marzo 2010, anziché dal 15 ottobre 2009 al 15 aprile 2010. In tale modo, si evita la chiusura in concomitanza delle festività pasquali 2010, così come richiesto dagli enti locali e dalle associazioni di categoria nel tavolo di coordinamento istituito presso l'ufficio della Protezione civile della sede prefettizia di Napoli. In caso di mancata conferma ovvero di decisione per un'ulteriore riduzione temporale delle finestre, si determinerebbe necessariamente una rimodulazione di tutte le attività lavorative e conseguentemente un allungamento dei tempi di ultimazione dell'opera. Va ancora ricordato che è stato istituito presso l'ufficio della Protezione civile della sede prefettizia di Napoli un tavolo di coordinamento cui partecipano gli enti locali e le associazioni di categoria. Per quanto concerne invece l'opportunità del potenziamento delle vie di collegamento marittimo, fermo restando l'impegno del Ministero delle infrastrutture e trasporti ad incrementare le cosiddette autostrade del mare, le competenze sui collegamenti marittimi della costiera amalfitana, come noto, spettano in via esclusiva alla Regione Campania.

devo rappresentare l'esigenza che questo programma, che è stato concordato in sede prefettizia e con tutti i soggetti e le associazioni interessati, non subisca alcun rallentamento.

essere interrotto il corso dei lavori per la riapertura della galleria, essendo la Penisola sorrentina oggetto di un flusso turistico proprio durante la settimana santa. C'è l'impegno e la determinazione di tutti a completare questi lavori nei tempi previsti, nella consapevolezza che questa struttura è fondamentale per l'economia turistica della zona

nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali" (1167) Derivante